«Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dell’istruzione, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero on. Anna ASCANI. Con viva cordialità, f.to Giuseppe CONTE».

legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato attribuito il il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero onorevole dott.ssa Emanuela Claudia DEL RE e signora Marina SERENI.

al disastro ferroviario che abbiamo potuto vedere anche sui media nazionali. Sono qui, oggi, a rappresentare

44 fronti di fuoco nella nottata tra il 29 e il 30 agosto nella sola Sicilia occidentale hanno devastato migliaia di ettari boschivi, deturpandone deturpandone le bellezze naturali e paesaggistiche, oltre ad arrecare ingenti danni alle persone e alle loro cose. Voglio fare solo alcuni nomi delle località più note: San Vito Lo Capo; la riserva naturale orientata dello Zingaro; Alcamo; sulle Madonie, il parco archeologico di Himera; Monte Iato e, per finire, il secolare bosco della Moarda, vanto e orgoglio del Comune di Altofonte, che sorge ai suoi piedi, e dove per poco non si è sfiorata la tragedia. Gente esperta dei luoghi, conoscitrice delle leggi del fuoco e sicuramente senza scrupoli, ha approfittato del caldo vento di scirocco per attuare questo piano criminale. Ora è facile indignarsi e imprecare contro coloro che materialmente hanno realizzato tale disastro. E questo l’ha fatto la gente comune, ma non può farlo chi è preposto a governare e a gestire quel territorio e le risorse umane di cui dispone per prevenire e valorizzarlo. Quando, poi, Quando, poi, la politica regionale vuole sfuggire alle proprie responsabilità, sovrapponendo l’emergenza degli sbarchi a Lampedusa, e fa la voce grossa con il Governo nazionale per celare le proprie inadempienze, nella speranza di stornare l’attenzione dell’opinione pubblica, ciò risulta a dir poco ridicolo, se non proprio grottesco. è in corso a Palazzo d’Orléans, sede del Governo regionale siciliano, una riunione della Giunta regionale per parlare delle misure di prevenzione da mettere in pratica contro gli incendi. Mi auguro che almeno questa volta una Giunta regionale sappia risolvere finalmente l’annosa questione forestale siciliana, che interessa più di 20.000 operai forestali impiegati a tempo determinato, alcuni per 151 giornate lavorative, altri per 101, altri ancora addirittura per 68.

20.000 unità dovremmo essere il fiore all’occhiello dell’intera Penisola italiana, dato che assorbiamo da soli più del 50 per cento degli impiegati nel settore a livello nazionale. E invece non è così: siamo tra i primi posti per numero di incendi e di superficie bruciata, e ciò non è gratis, perché comporta una grande spesa, che già la Corte dei conti ha quantificato, ordinando alla Regione una riforma organica, che tarda a venire, perché fa comodo lasciare le cose così STENOGRAFICO 1° Settembre 2020 Il Governo Musumeci si trova pertanto a dover rispondere a una procedura d’infrazione avviata già nel luglio 2019 dalla Commissione europea per aver abusato dei contratti a tempo determinato, in particolare dei lavoratori forestali, che lo stesso Musumeci ha più volte dichiarato essere tra le sue priorità. Mi auguro che a Palazzo d’Orléans si parli anche di dare dignità ai forestali attraverso un lavoro vero, che ne valorizzi le professionalità maturate nel tempo, e si smetta di ergersi a paladini dei siciliani contro un’invasione avvenuta più di mille anni fa, che ha portato alla nascita di una delle più belle espressioni culturali, concretizzata nell’arte arabo-normanna, oggi patrimonio dell’UNESCO.

la discussione sul tema scuola e istruzione. Ogni rappresentante politico del Parlamento italiano ha dimostrato sensibilità sull’argomento, che però non si è concretizzata in una proficua collaborazione. Molta attenzione è stata manifestata dal capo politico di Fratelli d’Italia quando il 19 aprile invitato il Governo a valutare la possibilità di riaprire il prima possibile le scuole per i bambini dai sei ai dodici anni. Ancora Fratelli d’Italia, il 6 agosto, dopo aver individuato criticità nei confronti del distanziamento sociale e delle classi pollaio,

con le rotelle, l’opposizione alza il polverone mediatico al limite dell’indecenza, al punto che una deputata ha accusato il ministro Azzolina di sperperare i soldi. Siamo arrivati alla bagarre delle rotelle, invece di pensare a costruire il futuro dei nostri figli: alla faccia del senso di responsabilità! Mi chiedo se finanziare la scuola pubblica e investire nel futuro del Paese equivalga per la minoranza a sperperare denaro. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre lavorato contro la dispersione scolastica, preservando il diritto allo studio dei nostri figli. Mai come con questo Governo la scuola ha visto tanti soldi investiti in pochi mesi (circa 7 miliardi da gennaio ad oggi). Tra i vari interventi, ricordo i finanziamenti all’edilizia scolastica, proprio come chiesto da Fratelli d’Italia; l’assunzione di nuovo personale tramite gli uffici scolastici regionali e, a brevissimo, due maxi concorsi; gli aiuti per l’acquisto di kit scolastici per le famiglie più bisognose, la digitalizzazione e la messa in sicurezza delle scuole. Vista l’anomala agitazione dimostrata negli ultimi giorni dal partito Fratelli d’Italia, viene da pensare che forse il problema non è che il Ministro

Vi chiedo se sia normale che il capo politico di un partito, donna e madre, possa giocare su un tema così delicato come il futuro dei nostri figli. Non si può cambiare bandiera a distanza di qualche mese. Quello che serve ora, onorevoli colleghi, è responsabilità e onestà intellettuale, soprattutto in un momento di grande fragilità emotiva per le famiglie italiane. Evidentemente, per le opposizioni fare terrorismo politico e creare panico rappresenta un’opportunità d’incremento dei consensi nei sondaggi, a discapito - ahimè

l’uso delle mascherine fornite dalla scuola, insieme al gel sanificante, e non ci sarà il plexiglass, come erroneamente racconta la destra italiana. La riapertura delle scuole per i nostri ragazzi è sinonimo di ripartenza, di normalità e di ripresa della socialità e dell’apprendimento in tutta sicurezza. (Applausi).